La seduta è aperta

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Grazie con condanne che prevedono anche l'interdizione, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e, ovviamente, la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

l'uso improprio di questo strumento di incentivazione ha procurato all'Italia più di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Il Governo Prodi aveva chiuso questa pagina non proprio edificante ammettendo a beneficiare di tali incentivi in via derogatoria soltanto due o tre impianti della Campania, cioè della Regione investita nel modo più drammatico dall'emergenza rifiuti. Con questo secondo decreto del Governo Berlusconi sull'emergenza rifiuti in Campania, invece, l'uso improprio del CIP6 viene di nuovo esteso. In particolare, viene massicciamente esteso ad una regione italiana - la regione

di chiudere la pagina dell'uso improprio dei CIP6. Se il Parlamento ed il Governo lo ritengono, si discuta di un incentivo specifico alla termovalorizzazione dei rifiuti, ma non si chiami incentivo alle rinnovabili qualcosa che serve per tutt'altro scopo.

e sugli ordini del giorno

che pensavamo definitivamente chiusa nel nostro Paese e cioè lo scandalo di finanziare con fondi che dovrebbero essere dedicati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili elettrica da fonti rinnovabili la produzione di energia elettrica da fonti che rinnovabili non sono. Si tratta di un onere rilevantissimo per le tasche degli italiani. Spesso, colleghi della maggioranza, affermate che non si mettono le mani nelle tasche degli italiani, ma in questo caso le state mettendo robustamente. L'anno scorso i cosiddetti contributi CIP6 sono costati sulla bolletta elettrica oltre 3 miliardi e mezzo di euro ai cittadini italiani e quando la vicenda del CIP6 sarà conclusa gli italiani avranno pagato più di 40 miliardi di euro di costi in più sulla bolletta elettrica. Questo è davvero uno scandalo su una questione che era stata chiusa e che adesso, in qualche modo, si riapre. Ricordo che sul totale della produzione di energia elettrica italiana

Ai colleghi della Lega che si stanno battendo per l'attuazione del federalismo nel nostro Paese - e noi stiamo lavorando perché questo si possa realizzare - chiedo cosa ha a che fare con il federalismo il fatto che tutti i cittadini italiani devono pagare più cara l'energia elettrica per finanziare quattro inceneritori in Sicilia. Noi, nei nostri territori, gli inceneritori li abbiamo realizzati facendoli pagare ai cittadini del nostro territorio. In base a cosa continuate a parlare di federalismo, se poi nella legislazione legislazione quotidiana questi principi vengono rinnegati? I cittadini italiani pagheranno più cara l'energia per finanziare l'incapacità delle amministrazioni territoriali di risolvere i loro problemi.

Grazie,

anzitutto al Governo, per coerenza, di restituire alla Protezione civile i fondi sottratti con la legge finanziaria per il 2009, senza i quali la prevenzione dei rischi sarà un esercizio impossibile.

Il comma 4 dell'articolo 2, ad esempio, affida al Sottosegretario la progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia, individuando a tal fine, previo parere degli enti locali, un sito idoneo in Campania, senza prevedere forme di collaborazione da parte della Regione interessata, tanto meno dagli enti locali interessati. Voglio ricordare all'Assemblea che le milioni di ecoballe stoccate in siti inappropriati non sono CDR, non sono cioè combustibile da rifiuti. Allora, si dà la possibilità al Sottosegretario di individuare un sito per mettere un altro termovalorizzatore per bruciare non si sa che cosa, ma quelle quelle balle non possono essere bruciate perché non sono frazione secca, c'è umido. Altrettanto si dica per il piano sugli inceneritori di cui all'articolo 9,

Vi sono, inoltre, diversi problemi rispetto alla normativa comunitaria. Lo strumento dell'ordinanza dì protezione civile ha incontrato più volte, in materia di appalti e affidamento di servizi, le censure della Commissione europea. È giusto e logico derogare, in situazioni emergenziali, a norme che rallenterebbero gli interventi rendendoli inefficaci. Ma le deroghe non dovrebbero mai travalicare i principi fondamentali delle direttive comunitarie. Si segnalano, a tale proposito, l'articolo 2, che introduce alcune deroghe alla disciplina di rimozione e trasporto dei rifiuti, anche pericolosi, nonché la lettera *c)* dell'articolo 9, che ammette all'incentivo per le fonti rinnovabili anche la parte non organica dei rifiuti. A tale proposito, seppur la deroga si limita agli impianti ammessi ad accedere agli incentivi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata prima del 2007, essa si trova letteralmente in contrasto con l'articolo 2 della direttiva quadro sulle fonti rinnovabili. La conseguenza potrebbe essere una procedura di infrazione che rallenterà, anziché accelerare, le opere che si intende velocizzare, accrescendo l'incertezza degli operatori per i finanziamenti sui quali si può davvero contare. Non solo, si riaprirà forse una procedura sulle cosiddette assimilate che era stata chiusa grazie alla norma che ora si modifica, ingannando di fatto le autorità comunitarie e finendo con l'arrecare danno a quanti, beneficiando degli incentivi, potevano contare su un quadro normativo certo e definito, ora rimesso in discussione. E' quindi davvero molto dubbia la piena compatibilità dell'articolo 9 con la normativa comunitaria delle disposizioni relative alla concessione di incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili. La scelta di modificare, per la terza volta in tre anni, il regime degli incentivi la platea dei beneficiari accresce l'incertezza del diritto e pone più problemi di quanti non ne risolva: accresce il contenzioso e aggira per via legislativa il dovere del Governo di indicare, con decreto ministeriale, gli impianti incentivabili. In tal modo, è chiaro, chi si sentirà leso in un interesse legittimo non potrà fare ricorso al giudice amministrativo. Se è davvero necessario incentivare taluni impianti, e potrebbe esserlo, si abbia il coraggio di farlo con fondi a ciò specificamente dedicati, senza incidere sulla quota destinata alle autentiche fonti rinnovabili (pensiamo al solare termodinamico o a concentrazione). Soprattutto, si eviti di farlo surrettiziamente ed a spese dei cittadini che pagano la tariffa elettrica e la componente a ciò dedicata. Siano quindi destinate risorse *ad hoc* e si affronti apertamente un dibattito in Parlamento: non mancheranno, da parte delle opposizioni, suggerimenti e proposte come sono venute anche in questi giorni sul decreto. Su tutti questi articoli sono stati presentati appositi emendamenti migliorativi e correttivi. E' stato inoltre presentato un emendamento, che venne erroneamente e ingiustamente giudicato microsettoriale e localistico in finanziaria (quando invece reca lo stesso ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 6 che il Governo giudica, al contrario, generali ed astratte!) volto ad assicurare una prioritaria attenzione alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti occupati da depositi temporanei di rifiuti in aree dove vige lo stato di emergenza, ed oggi, per fortuna, il Sottosegretario ha accolto una raccomandazione in tal senso. In Campania, nello specifico, il problema ambientale riguarda i luoghi dove sono state depositate le cosiddette ecoballe. Si tratta di un problema assai grave, in particolare per alcune località interessate da anni da questa emergenza, che merita di essere preso in considerazione nonostante l'imminente scadenza del decreto-legge in esame. I fondi per le bonifiche esistono, esiste la struttura e le leggi per attuarle. Si tratta di avviarle effettivamente o, in alternativa, di garantire una priorità a questi interventi.

toglierci qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del sindaco di Napoli, la signora Iervolino. A Napoli, quasi fossimo in una commedia di De Filippo, la realtà si è trasformata in farsa: un sindaco che ha visto accumularsi montagne di rifiuti in ogni angolo della città non ha avuto il buon senso di trarre le dovute conclusioni ed andarsene. È, al contrario, rimasto e rimane al suo posto, come un mozzo qualsiasi che per sopravvivere alla tempesta si limita a legarsi all'albero maestro della nave, sperando che non affondi. Come se non bastasse, l'abbiamo sentita, in piena emergenza, anche sanitaria, fare spallucce dichiarando, con tono scocciato: «Ma cosa volete che sia? Non sta morendo nessuno». È con questi atteggiamenti che ha offeso anche il popolo napoletano, dopo averlo umiliato e mal governato, facendogli, per causa sua, subire addirittura leggi speciali, talvolta davvero stringenti, ma, come ben sappiamo, necessarie ad arrestare il degrado causato da negligenze di una classe dirigente inadatta, inetta e incapace perfino di gestire l'ordinaria amministrazione. Se il Sindaco continua ad avere il cattivo gusto di rimanere sul suo scranno, facendo credere che la decenza non ha più cittadinanza a Napoli, ricordo che potrebbe essere rimosso, anche senza questo decreto, perché l'articolo 142, primo comma, del decreto «Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico». Credo che nella vicenda dei rifiuti in Campania di motivi ce ne sono da vendere. Non saremo certo noi a chiedere al ministro Roberto Maroni di prendere tale decisione, nel rispetto dei principi autonomisti che da sempre ci animano. Ma, cara Rosetta, vorrei ricordare un episodio:

il decreto di sospensione in attesa di rimozione da sindaco di Lazzate, ordinato proprio dal Ministro dell'interno. Fui sospeso, e la colpa era di aver difeso i miei cittadini, la mia gente e la comunità che rappresentavo. Fui sospeso perché avevo compiuto fino in fondo il mio dovere nell'interesse dei miei cittadini. Fu un attacco non solo a me, ma a tutta la Lega Nord. Fu in quel momento che entrò in gioco una forza che a lei, cara Rosetta, davvero manca, la forza della gente: tutti i lazzatesi e decine di migliaia di simpatizzanti della Lega Nord scesero in piazza per difendere un sindaco che aveva fatto il proprio dovere. Tutti si schierarono contro la decisione di un Ministro, che arrivò perfino alla menzogna in un *question time* alla Camera, in diretta televisiva, per difendere le sue posizioni. Noi vincemmo la battaglia, io fui reintegrato al mio posto di sindaco, ma il bello di questa storia è che il Ministro dell'interno era lei, signora Rosa Russo Iervolino. Era lei che sospendeva i sindaci contro la volontà popolare, ma oggi, in sua difesa, nessun cittadino sfilerebbe per le vie di Napoli; in sua difesa nemmeno un sostenitore del suo partito scenderebbe in piazza, perché è ormai diventata un peso, non solo per Napoli, ma anche per i suoi compagni politici. Cara Rosetta, sono passati quasi dieci anni da quella da quella mattina; qualcuno li chiamerebbe ricorsi storici, per noi hanno il sapore della giustizia. Infatti, ora sono io e la Lega Nord ad inviarle un bel foglio di via, senza Carabinieri, senza carte bollate, diciamo che è un invito, ma gridando in quest'Aula, anche a nome dei suoi concittadini napoletani, oggi mettiamo i sigilli al suo fallimento politico-istituzionale; faccia le valigie e se ne vada a casa!*(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).* E, mentre se ne va dal suo ufficio, perda cinque minuti per raggiungere Via Santa Lucia 81, sede della Regione Campania, prenda a braccetto il suo compagno di partito Antonio Bassolino e che Dio vi perdoni. Sono un cattolico e come tale sono portato al perdono, ma il perdono tiene vivo il ricordo.

il Partito Democratico sente per intero la responsabilità di contribuire all'uscita dal tunnel dell'emergenza rifiuti in Campania e che di tale responsabilità intendevamo farci carico davanti ai cittadini campani e davanti a tutta l'opinione pubblica. di condividere la scelta di Guido Bertolaso come guida non solo tecnica della gestione dell'emergenza. Per questo allora ci astenemmo, pur sottolineando tutti i rischi di un eccesso di deroghe alla legislazione ordinaria, alla giurisdizione ordinaria, all'amministrazione ordinaria - presente in quel primo decreto. Oggi noi confermiamo quell'assunzione di responsabilità, che peraltro si è concretizzata in una piena collaborazione all'opera svolta da Bertolaso da parte del Partito Democratico in Campania. La confermiamo malgrado l'uso demagogico, propagandistico, da illusionisti più che da statisti, che il Governo e la maggioranza hanno fatto in questi mesi dell'emergenza e che è risuonato anche adesso nelle parole del senatore Monti; con il Presidente del Consiglio, l'ha ricordato nel suo intervento il senatore De Luca, che una volta alla settimana va a Napoli per proclamare che l'emergenza è finita sebbene le cose, come sanno benissimo anche i colleghi campani della maggioranza, stiano in modo molto diverso. Confermiamo quell'assunzione di responsabilità, ma vediamo decisamente ingigantiti tutti i motivi di preoccupazione e di critica di fronte a un decreto che in molte sue parti ci appare non condivisibile e che soprattutto sembra muovere non verso il ritorno all'ordinaria amministrazione, ma verso una sorta di normalizzazione della gestione eccezionale, derogatoria, verso l'idea che in Campania per gestire i rifiuti debbano valere stabilmente principi, diritti diversi da quelli che valgono altrove. L'articolo 6, quello che introduce solo per il territorio campano il reato di abbandono di rifiuti ingombranti, è l'emblema di questa impostazione inaccettabile. Il senatore Casson, illustrando la questione pregiudiziale posta dal nostro Gruppo, ha tratteggiato tutti gli elementi che fanno dubitare anche della costituzionalità di questa norma. Io aggiungo poco altro. Dico che noi naturalmente siamo d'accordo sull'esigenza di sanzionare più duramente comportamenti incivili e che recano un danno alla collettività, com'è abbandonare per la strada un frigorifero o un armadio. Ma le sanzioni più dure devono valere per tutti e dappertutto; devono distinguere tra rifiuti solo ingombranti e, faccio un esempio, rifiuti speciali; devono rispondere a un minimo criterio di proporzionalità tra gravità dell'illecito e gravità della pena. Ma che Paese è quello che avete in mente, nel quale se uno abbandona una vecchia cucina a Napoli rischia tre anni e mezzo di carcere e se l'abbandona a Campobasso o a Bergamo o a Roma rischia qualche centinaio di euro di multa? O nel quale la pena massima per chi abbandona rifiuti è superiore a quella minima per chi organizza traffico illecito di rifiuti industriali? Qualcuno nella maggioranza ha giustificato questa norma assurda sostenendo che rappresenta un deterrente all'abbandono di rifiuti per la strada. A me pare soprattutto un incentivo a caricarli in macchina e ad abbandonarli qualche centinaia di metri oltre il confine della Campania. In questo decreto-legge sono poi state inserite misure e norme che con l'emergenza rifiuti in Campania non hanno nulla a che fare e che in molti casi sono assai negative. Come la previsione, un po' bislacca e ipercentralista, di un piano nazionale degli inceneritori, in uno scenario legislativo nel quale, a parte il caso delle Regioni in emergenza, la gestione dei rifiuti e tutte le scelte connesse sono di competenza di Regioni ed enti locali. O come la norma che, per fare un favore a qualche azienda, autorizza l'utilizzo in casa del cosiddetto tritarifiuti, quell'aggeggio che si monta sotto il lavabo e tritura i rifiuti organici. Peccato che, come sa qualunque idraulico, nelle case italiane i tubi di scarico delle acque bianche, nel 95 per cento dei casi, non siano compatibili con questa straordinaria innovazione, che rischia di costare alle famiglie molto più di quanto farà guadagnare a chi commercializza i tritarifiuti. Altra norma aliena è quella che riguarda il cosiddetto CIP6, consentendo che in particolare i termovalorizzatori progettati in Sicilia possano beneficiare degli incentivi previsti per le rinnovabili. La questione del CIP6 è molto semplice: da anni in Italia gli utenti pagano in bolletta una somma notevole come contributo per lo sviluppo delle energie rinnovabili. In tutto - l'ha ricordato il senatore Giaretta - hanno pagato circa 40 miliardi di euro, ma tre quarti di questa somma enorme non è servita a incentivare le rinnovabili, bensì per finanziare la produzione di energia nei termovalorizzatori o nei cementifici. Il Governo Prodi aveva posto fine a questa vera e propria truffa, che peraltro ci ha procurato svariati richiami dall'Unione europea, ammettendo una deroga solo per tre impianti campani indispensabili per chiudere l'emergenza. Il Governo e la maggioranza, invece, hanno deciso di continuare con un uso improprio e truffaldino degli incentivi CIP6, soprattutto assegnando 2 miliardi di incentivi presi dai CIP6 alla Sicilia. Ora, non ne faccio una questione ideologica: se si ritiene che gli inceneritori debbano essere incentivati, lo si dica, si proponga una norma *ad hoc* e se ne discuta; non si può, però, continuare ad ingannare i cittadini, dicendo loro che i soldi che danno servono per l'energia solare, utilizzandoli invece per bruciare i rifiuti. La via da seguire è quella indicata dall'Europa, del resto prevista anche in questo decreto, al comma 1-*bis* dell'articolo 9: i rifiuti hanno diritto a beneficiare degli incentivi alle rinnovabili per la loro parte fatta di materia organica, cioè di materia per l'appunto rinnovabile che è circa la metà; per il resto, si chiuda una volta per tutte la storia ingloriosa dell'uso improprio degli incentivi CIP6. Nonostante alcuni aspetti condivisibili, che pure vi sono in questo provvedimento, in particolare l'articolo 3, nella versione corretta uscita dalla Camera, che fissa i criteri per il commissariamento dei Comuni e degli enti locali inadempienti sulla raccolta differenziata, tutto questo ci spinge a votare contro il decreto oggi in esame. Votiamo no e rivolgiamo un appello, in particolare al Governo: fermatevi su questo piano inclinato di deroghe, di eccezioni, di procedure sempre meno democratiche - sui rifiuti, come su altri temi importanti: penso al nucleare - e sempre più centraliste (si occupi di questo, senatore Monti, invece che delle piacevolezze che ci ha raccontato) e di processi legislativi sempre meno aperti al contributo del Parlamento. Votiamo no, colleghi, perché ci ribelliamo all'idea che solo militarizzando la Campania, riducendo i diritti dei campani e rinnegando principi irrinunciabili, come l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, sia possibile mettere fine a questa lunghissima notte dell'emergenza rifiuti.

*(PdL)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, signori colleghi senatori, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo PdL al provvedimento in esame, mi permetto di svolgere qualche breve riflessione conclusiva. Gli effetti positivi delle norme contenute in questo provvedimento ci hanno fatto dimenticare la difficile e drammatica situazione emergenziale che si è abbattuta sulla Campania nella primavera scorsa per quanto riguarda i rifiuti: una vera e propria catastrofe, che ha danneggiato non solo Napoli e la Campania, ma l'immagine dell'Italia intera. Sembra passato un secolo, da quando le emittenti televisive di tutto il mondo aprivano i notiziari con l'immagine dei cumuli di rifiuti incendiati per le strade e le scene di guerriglia dei contestatori (penso a Chiaiano, a Pianura e a Santa Maria La Fossa). L'Esecutivo appena insediatosi ha dovuto fronteggiare non un'emergenza, ma una vera e propria tragedia. La situazione è stata gestita dal Governo con la massima determinazione incisività e la dovuta intransigenza, dimostrando per la prima volta - voglio sottolinearlo - che lo Stato è presente per riaffermare che le assurde contestazioni di pochi non possono averla vinta sugli interessi generali del Paese. Ebbene, a pochi mesi dal primo Consiglio dei ministri tenutosi proprio nella città partenopea, il Governo non solo ha rimosso i rifiuti dalle strade di Napoli, ma ha avviato a soluzione la complessa problematica in tutta la Campania. Questo è stato possibile anche grazie alle misure adottate con il provvedimento che licenzieremo oggi, misure che presto porteranno la Campania in quella tanto auspicata normalità.

anniversario, e si fissa come termine per il rientro nella gestione ordinaria il 31 dicembre 2009. In questa chiave va letta anche la nomina a Sottosegretario di Stato dell'attuale direttore generale della Protezione civile dottor Bertolaso. Con il provvedimento che noi licenziamo oggi si prevedono la rimozione definitiva e la messa a dimora dei rifiuti indifferenziati e pericolosi si prevedono norme sanzionatorie, fino allo scioglimento, per i consigli comunali e provinciali che non rispettano gli obblighi posti a loro carico circa la programmazione ed organizzazione della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti. gli enti locali non collaboravano, anzi, intralciavano l'opera del commissariato nella individuazione dei siti per le discariche; oggi, invece, i comuni e le province si pongono con un nuovo protagonismo attivo. Si definiscono poi le modalità per l'affidamento del servizio di raccolta per i comuni della provincia di Caserta, prevedendo che le gare si svolgano sotto la vigilanza della prefettura che funge come una vera e propria stazione appaltante; viene definito anche il livello delle responsabilità e le sanzioni, anche penali, a carico di chi abbandona i rifiuti in modo incontrollato sul suolo pubblico o privato, ovvero li incendia. Riteniamo, infine, sia stato importante, utile ed opportuno inserire la norma di cui all'articolo 7, relativa alla campagna informativa, per coinvolgere e sensibilizzare l'opinione pubblica sul sistema di raccolta differenziata e la norma inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati di cui sulla formazione scolastica, affinché i giovani metabolizzino l'importanza di rispettare il territorio dove si vive e di preservare un ambiente sano. Riteniamo, in conclusione, che le misure adottate con questo provvedimento, che già stanno dando risultati soddisfacenti, accompagneranno la Campania verso una nuova fase di normalità e responsabilità. Per tutti questi motivi, voteremo

Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per la semplificazione normativa e dal Ministro della giustizia:* «Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa»

***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare***

di euro per la promozione del nostro olio di oliva extravergine. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva. Per le altre considerazioni mi rimetto

la senatrice Antezza.

Buora per aver condotto in modo magistrale i lavori, il relatore Piccioni e, ovviamente, anche il presidente Azzollini per l'aiuto che ci ha dato.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sugli articoli

ci sono però scadenze e risorse per affrontare l'immediato. Pertanto, preannuncio che il nostro sarà un voto di astensione, considerando che gran parte delle modifiche inserite è frutto del nostro lavoro e della nostra determinazione,

sulle due questioni principali del fondo di solidarietà e delle agevolazioni per gli oneri sociali per le zone svantaggiate, affinché sia migliorato ciò che oggi è assolutamente inadeguato. Signor Ministro, vedremo dove finisce la sua capacità di comunicazione e quel pizzico di demagogia che a volte rinveniamo nel suo operato, e dove inizia la concretezza delle scelte, perché oggi ancora non la vediamo.

da lei, signor Ministro, può essere considerato complessivamente positivo. Certamente non è risolutivo, ma lei lo sa meglio di noi: questo è un primo grande intervento, al quale ne seguiranno altri che lei, del resto, ha già annunciato.

quella dignità e anche quelle risposte in termini economico-finanziari che in questo momento sono veramente attese. Cari colleghi della Commissione agricoltura, credo che avremo molto da lavorare nel prossimo anno, insieme al Ministro e a tutti gli agricoltori italiani. Rivolgo un augurio a tutta l'agricoltura italiana e alla pesca.

ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 dell'articolo 32 le parole: "quanto ad euro 4.910.000 per l'anno 2010" siano sostituite dalle altre: "quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dall'anno 2010" e che al comma 2 del medesimo articolo le parole: "per l'anno 2010"

riguarda la cooperazione transfrontaliera, la lotta al terrorismo, alla criminalità e alla migrazione illegale e, inoltre, l'istituzione

**Il Senato non approva.**

Farò due premesse. Presso il Ministero è in atto un'attività di ricerca e di realizzazione di un sistema informatico che riguarderà l'intero comparto giudiziario: banche dati che dovranno comunicare Si tratta di una riforma iniziata con il vecchio Governo Prodi e che questo Governo, almeno nelle dichiarazioni del ministro Alfano, sta portando avanti, io dico, in maniera positiva. L'oggetto dell'attività è stato poi trasfuso in un disegno di legge, ora all'esame della 2a Commissione permanente, presentato dall'opposizione, ma che trova

che riguardano il DNA di persone indagate o imputate di crimini di altissimo livello offensivo. Si tratta di un materiale complessivamente di origine o di pertinenza giudiziaria.

abbia la vigilanza e, quindi, l'autorizzazione per ogni tipo di modifica e di trasformazione da parte dell'autorità giudiziaria, che viene individuata nel procuratore

deve essere appositamente selezionato, autorizzato e tenuto addirittura al segreto d'ufficio.

*(PdL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.500, ma ribadisco l'urgenza che il Governo si occupi delle problematiche legate all'istituzione della figura del garante dei diritti dei detenuti,

creazione di un soggetto interlocutore di natura istituzionale che possa porsi tra l'autorità penitenziaria e i detenuti. Tale soggetto già esiste in molte Regioni, in molti Comuni e in molte Province, ma è privo di qualsiasi tipo di disciplina,

dichiarazione di voto. Grazie, signora Presidente.

che hanno ritenuto opportuno convergere sulla utilizzazione di una serie di strumenti (tra cui la banca dati del DNA e lo scambio di informazioni) e lo e lo hanno fatto per dare un impulso ad una lotta che non può che essere europea non solo al terrorismo, ma anche alla immigrazione clandestina e a quelle forme di criminalità transnazionale

al Ministro dell'interno del tempo, Amato, di aver manifestato l'intenzione di aderire a questo trattato, ancorché non abbia avuto la forza politica nella passata legislatura per consentirne la ratifica. ratifica. Credo che dovremmo andare avanti su questa strada perché il tema dell'immigrazione clandestina deve essere affrontato a livello europeo. Laddove non si riesca a farlo con le regole previste dal Trattato dell'Unione per i veti incrociati tra i vari Paesi, credo che questa strada, segnata dal Trattato di Prum, sia un buon viatico. E su questo il nostro Paese deve assumere una iniziativa forte. Per queste ragioni, votiamo convintamente a favore di questo provvedimento e diamo atto al sottosegretario Mantovano dell'impegno profuso per portarlo a compimento.

che peraltro - ed era quello che avevo messo in evidenza in sede di discussione generale - non ha fatto altro che utilizzare il lavoro svolto nella scorsa legislatura e che non fu portato a compimento a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, ma il disegno di legge era già stato presentato ed io avevo coordinato i lavori della commissione ministeriale.

capo dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, presidente Gianfranco Manzo, che insieme alle forze di polizia, ai carabinieri ed ai reparti speciali del RIS e della polizia scientifica collaborò per Grazie. indubbiamente faciliterà il lavoro degli inquirenti e della magistratura nell'interesse cittadini. Non era quindi polemico il mio

lavoro svolto. Rivendicare il buon risultato del proprio lavoro non penso abbia una connotazione polemica. Questo è il risultato anche del mio lavoro.

che è stato importantissimo per questo e per molti altri disegni di legge, che la maggioranza ed il Governo continuano a ricopiare, che sono stati presentati dal nostro Gruppo e dal Gruppo del Partito Democratico. Quindi, non c'è nulla di polemico non c'è una primogenitura, c'è soltanto la rivendicazione del buon lavoro svolto, che ci mette in linea con gli altri Stati europei e che dota il nostro Paese di un ottimo strumento investigativo. Ovviamente

con oltre 2 milioni di profili. È chiaro che per noi ci vorranno anni per arrivare a tali risultati, però ci siamo avviati lungo questa strada e abbiamo dotato le nostre forze di polizia, che sono considerate ad un livello di eccellenza mondiale, di un ulteriore strumento di contrasto alla criminalità. Il nostro voto sarà quindi favorevole e ringrazio il Parlamento, la Commissione, i relatori ed anche il Governo per aver condiviso il nostro lavoro ed averlo portato a conclusione. Presidente, colleghi, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo provvedimento, per noi estremamente importante, perché rappresenta l'attuazione del pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri a maggio 2008. Di quel pacchetto sicurezza ormai sono in vigore tutti i tutti i provvedimenti. Con questo voto completiamo l'opera; rimane il disegno di legge n. 733, che verrà discusso in Aula a gennaio, alla ripresa dei lavori. Finalmente possiamo dire con orgoglio che abbiamo un Governo e soprattutto un Ministro dell'interno che sa governare il tema della sicurezza, sa dare risposte concrete ai nostri cittadini. Quindi, con orgoglio voteremo a favore di questo importante provvedimento.

frutto di una convergenza estremamente positiva. Vorrei ringraziare il senatore Casson, i colleghi del Gruppo del Partito Democratico e quelli degli altri Gruppi, che hanno dato un contributo prezioso per migliorare il provvedimento che stiamo per votare. Sottolineo con soddisfazione che il Capo IV,

del DNA e il suo laboratorio centrale. L'adesione poi al Trattato di Prum, per contrastare criminalità, terrorismo e migrazioni illegali, è una misura di cooperazione fondamentale per il nostro Paese e l'Europa. La mia conclusione è la seguente, Presidente: su questa materia, che esige la collaborazione tra maggioranza e opposizione, quando si registra la volontà di collaborare penso che facciamo il nostro dovere. Apprezzerei in questo caso che anche i colleghi della maggioranza e il Governo facessero notare la qualità e l'utilità di questa convergenza, che non sempre si registra. In questo caso si è registrata: decine di proposte dell'opposizione sono state recepite e integrano un testo che ha un grande valore. Penso che ciò dovrebbe avvenire sempre sempre - quando sono in questione esigenze di sicurezza nazionale, decisioni che riguardano le libertà fondamentali e i diritti dei cittadini

che si batte per le sue idee, che propone e che contribuisce a costruire le soluzioni nell'interesse generale. *(Applausi Signor Presidente, l'Italia era il penultimo Paese che doveva ratificare il Trattato di Prum; lo abbiamo fatto in sette mesi, in sette mesi, a seguito di altri provvedimenti, come il decreto-legge n. 92 del maggio scorso e la quasi approvazione dell'Atto Senato n. 733. Questa è la politica dei fatti della

con cui il nostro Paese riesce a realizzare il secondo pilastro delle politiche di sicurezza dell'Unione europea. È uno strumento indispensabile per il coordinamento dell'attività antiterroristica e di contrasto ai più gravi fenomeni della criminalità

la Commissione bilancio, che ha permesso, come sempre con ampia collaborazione, di coprire finanziariamente questo provvedimento. Non posso che condividere l'appello a che su questioni che incidono sulla sicurezza quotidiana dei cittadini ci sia il massimo della convergenza, così come è stato sottolineato prima in quest'Aula.

negli Stati Uniti della ratifica e l'entrata in vigore del Protocollo.